uno dei provvedimenti che - non lo nascondo - crea qualche imbarazzo, ma lo voteremo per le conseguenze che si verrebbero a creare se tale norma, già approvata dalla Camera, non incontrasse l'espressione di un voto favorevole da parte di quest'Assemblea. Ricostruisco brevemente le cause che hanno determinato la necessità del decreto-legge di proroga. Il 30 ottobre è scaduto il termine previsto per l'adeguamento delle prescrizioni sugli impianti soggetti a tale disciplina, recependo la direttiva 96/61/CE dell'Unione Europea, Europea, che introduceva l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per attività produttive quali: quelle energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerari, industria chimica, gestione dei rifiuti, allevamento degli animali, vetrerie, cartiere, cementifici, raffinerie e macelli. Tale autorizzazione, indirizzata alle attività industriali sopra citate, siano esse esistenti, nuove o sostanzialmente modificate, doveva includere valori limite di emissione basati sulle migliori tecniche disponibili al fine di implementare un approccio integrato contro le emissioni industriali nell'aria, nell'acqua, nel suolo. Dal 1996, anno di emissione della direttiva europea, l'Italia recepisce la direttiva stessa solo nel 2005,

Il differimento è dovuto al fatto che, a tutt'oggi, nessuna delle autorità competenti (le Regioni per l'80 per cento, lo Stato per il 20 per cento) ha concluso i procedimenti pendenti delle oltre 8.000 aziende, nonostante le domande da parte delle imprese siano pervenute nei tempi previsti e con relativi fondi impiegati.

risultano connessi anche alla mancata approvazione, da parte delle Regioni, dei piani per la qualità dell'aria. Pertanto, il differimento del termine che qui si propone si rende necessario per evitare possibili cessazioni delle attività produttive in questione e sanzioni amministrative e penali. Infatti, in assenza del citato differimento si verrebbe a creare, anche sotto il profilo sanzionatorio, in base all'articolo 16, la situazione per la quale chi esercita una delle attività soggette ad AIA senza la suddetta autorizzazione è soggetto alla sanzione penale dell'arresto fino ad un anno e ad un'ulteriore ammenda. La proposta che viene avanzata fissa un termine ultimo per la presentazione delle domande al 31 marzo 2008 e, viste le procedure farraginose contenute nel dispositivo, si provvede anche, all'articolo 2, comma 1-*ter*, ad adottare poteri sostitutivi da parte del del Ministero nei confronti delle Regioni che non dovessero attrezzarsi per il disbrigo delle domande. È evidente che, in questo caso, i poteri sostitutivi dovranno essere attribuiti al più presto. Inoltre, all'articolo 2-*ter* si invita il Governo a presentare al più presto una relazione in ordine allo stato di attuazione di questa normativa.

ha approfondito molto la questione. Pertanto, si ritiene che il termine che qui si propone possa servire ad evitare procedure di infrazione, dia risposte immediate

che, per responsabilità delle amministrazioni centrali e anche periferiche dello Stato, non sono state emanate in risposta alle oltre 8.000 domande che sono state presentate.

A questo punto, sono migliaia le situazioni che rischiano di andare fuori legge e di incorrere quindi nelle sanzioni amministrative e penali che sono previste. Laproposta del Governo di posticipare al 31 marzo 2008 la data di scadenza delle autorizzazioni è senz'altro da accogliere e da sostenere. Certamente questa dovrà essere accompagnata però da alcuni da alcuni impegni che il Governo deve assumere in prima persona per non ricadere in analoga situazione alla scadenza del 31 marzo 2008. In particolare, dovranno essere agevolate tutte le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti che sono state regolarmente presentate entro i termini previsti e i cui gestori possono dimostrare di aver assicurato in ogni passaggio, come previsto dalla direttiva europea, l'adeguamento alla normativa europea e si possa in questo caso rilasciare un'autorizzazione sulla base di un'autocertificazione su cui le competenti autorità nazionali potranno successivamente intervenire per controllare. Credo che questo impegno il Governo dovrà assumerlo in modo categorico per non cadere anche e soprattutto in una sanzione che l'Unione Europea altrimenti sarà costretta ad infliggere al nostro Paese. come ha giustamente rilevato anche la relatrice, che ha presentato un apposito ordine del giorno, allo scopo di contribuire al raggiungimento degli stessi obiettivi di qualità dell'aria che scattano dal 1° gennaio 2008, è importante che il rilascio del provvedimento di esenzione, che è stato richiesto da molte aziende, sia effettivamente rilasciato dalle autorità centrali, tenuto conto che queste aziende si sono impegnate ad applicare le migliori tecnologie per limitare l'inquinamento dell'aria. Infine, per i nuovi impianti che hanno ottenuto la compatibilità ambientale e sono oramai in fase avanzata di costruzione, è giusto dare un'autorizzazione provvisoria per poter effettivamente smaltire il numero più alto possibile di domande alla scadenza del 31 marzo 2008. Con questi impegni che raccomandiamo al Governo, sosteniamo il provvedimento Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che ci accingiamo purtroppo a convertire è un decreto-legge che si configura necessario per non far chiudere oltre 8.000 imprese italiane di rilievo, come raffinerie, industrie chimiche e cartiere. Sottolineo "purtroppo" perché è un decreto-legge che certamente non servirà a risolvere i problemi e alla scadenza prevista sarà necessario concedere una nuova proroga e al tempo stesso mettere necessariamente in preventivo il fatto che verosimilmente sarà aperta dall'Unione Europea una procedura di infrazione. Il problema, onorevoli colleghi, non è legato a ritardi nell'assolvimento degli adempimenti che facevano carico alle imprese italiane, ma al fatto che la pubblica amministrazione e segnatamente il Ministero dell'ambiente, attraverso una cancellazione per ragioni meramente politiche della commissione per la valutazione dell'impatto ambientale nominata dal precedente Governo, con conseguenti mesi e mesi di assoluta inattività istruttoria in attesa della nomina della nuova commissione, non ha ancora concluso tutti i procedimenti pendenti, nonostante le imprese abbiano già tempestivamente presentato le relative domande e assolto ai conseguenti oneri. Questo è il vero problema al nostro Certo, vi è la necessità di un provvedimento che consenta ad imprese di tale importanza per l'economia del Paese di continuare a lavorare, però è del tutto incongruo porre una nuova scadenza al 31 marzo 2008 per due motivi. Da un lato, è certamente improbabile che ciò che non si è fatto in due anni si riesca a fare in cinque mesi, a prescindere dal fatto che sia stato previsto un potere sostitutivo che però, di fronte alla mole di pratiche che si è andata accumulando, sembra francamente - *absit iniuria verbis* - un pannicello caldo; dall'altro, dare una scadenza comunque diversa rispetto a quella del 30 ottobre 2007, secondo quanto previsto dall'Unione Europea, sarà sicuramente fonte di una messa in mora del nostro Paese e dell'avvio di una conseguente procedura di infrazione. È l'anello debole di questo provvedimento, che voteremo, con grande disagio, solo perché le imprese italiane non siano ulteriormente penalizzate

per permettere la prosecuzione dell'attività produttiva di oltre 8.000 industrie basilari (come raffinerie, industrie chimiche, cartiere), mantenere l'impianto normativo del solo articolo 2,

Con questo spirito ci accingiamo a votare il decreto in esame: lo facciamo perché le nostre imprese non paghino un ulteriore prezzo a fronte della vostra politica, anche se resta indubbio dell'ennesima dimostrazione di un atteggiamento miope che va contro gli interessi veri della Nazione.

le esigenze della macchina ormai incancrenita dell'organizzazione territoriale dello Stato decentrato. Il nostro voto, lo ripeto,

Il nostro Ministero dell'ambiente non produce più un atto. Oltre ad aver bloccato, per decisione puramente politica, gran parte delle infrastrutture più importanti per il Paese per restare nel contesto europeo, costringe i nostri imprenditori a non poter ottenere le necessarie autorizzazioni per portare avanti il loro lavoro. In questo giorni stiamo vedendo - è sotto gli occhi di tutti - lo sfascio in cui si trova il Paese grazie all'operato del Governo. È un tassello che si aggiunge di incertezza, precarietà e non corrispondenza alle direttive europee grazie esclusivamente a questo Governo. Ormai da un anno e mezzo il Ministero dell'ambiente non governa più l'Italia e nel decreto in esame si chiede anche l'attivazione di un potere sostitutivo, senza indicarne peraltro le modalità

modelli di efficienza, ma è altrettanto vero che tutto dipende dalla testa. Il Ministero dell'ambiente sta dimostrando la sua assoluta incapacità di risolvere questi problemi. Ha creato solamente confusione normativa volendo, per motivi politici, interrompere le attuazioni dei decreti legislativi varati dal precedente Governo senza saperle sostituire con con modalità e prescrizioni altrettanto efficienti e valide, per cui ci troviamo in una situazione di stallo assoluto. Come ha detto il collega Leoni, siamo certi che entro il 31 marzo 2008 questo problema non si potrà risolvere. Forse ci troveremo dinanzi ad un'altra proposta ad un'altra proposta di proroga e non so con quali modalità, perché - come tutti sappiamo - la reitera dei decreti in sede costituzionale è oramai prassi non più avallabile. Quindi non sappiamo Chiedo al Governo e al relatore se già in questa sede non ritengano di dover proporre un termine più congruo. La nostra partecipazione al voto di questo provvedimento

direttiva comunitaria. In questa sede chiedo al Governo e alla relatrice se non siano dell'idea di proporre un termine più ampio con un passaggio velocissimo alla Camera, che sarà sicuramente accolto, così da dare una prospettiva di maggiore serenità ai nostri imprenditori e al Governo stesso nell'emanazione dei provvedimenti necessari. Le commissioni nazionali non sono ancora state completamente definite. I decreti di rinomina, voluti dal Ministro per ribaltare la situazione

nell'emergenza non possiamo sottrarci a concedere la proroga, ma noi la riteniamo assolutamente inefficace. Non aggiungo altro, perché lo sfascio del Ministero dell'ambiente è sotto gli occhi di tutti noi componenti della Commissione, ma soprattutto dei cittadini,

Signor Presidente, illustri senatrici e senatori, il provvedimento giunge a conclusione di un *iter* particolarmente tormentato.

straordinario per consentire al nostro Paese di allinearsi alle normative europee. Sono dieci anni che questa direttiva stenta a decollare tra diverse responsabilità. Oggi occorre forse tornare sulla questione del rapporto tra centralismo e decentramento, dato che i limiti riguardano entrambi. Non si può affermare, tuttavia, che non abbia funzionato la sola istituzione centrale. Certo, vi sono nostri limiti ma anche limiti delle Regioni. Dico questo non tanto per invocare

Il Governo si accinge, nonostante la ristrettezza dei tempi, a svolgere fino in fondo la sua parte, sapendo che i tempi sono strettissimi. Per questo credo sia più che opportuna una collaborazione

di concerto con il Ministro per le politiche europee. Credo che sia questo un segno di responsabilità che il Governo ed il Ministero dell'ambiente, in questo momento, si assumono per creare le condizioni idonee affinché si possa definire questa problematica in maniera corretta così come da troppo tempo viene invocato dagli imprenditori e non solo da questi. Ringrazio, pertanto,

Signor Presidente, il Gruppo Verdi-Comunisti Italiani voterà a favore del disegno di legge di conversione del decreto-legge

La norma transitoria è volta a consentire la prosecuzione dell'attività, se è stata presentata la domanda nei termini; questa è anche una garanzia che tale attività venga svolta nel rispetto della normativa vigente. Dopo tale proroga ci

al Ministero dell'ambiente, quest'ultimo deve emanare immediatamente i decreti per stabilire le tariffe a carico dei richiedenti l'autorizzazione integrata ambientale; soprattutto, in questo impegno è fondamentale disporre una ricognizione dettagliata

vicenda delle competenze tra Stato e Regioni auspico con sincerità, così come su altre questioni di grande rilevanza per l'ambiente, una riflessione più articolata e maggiore cautela quando invochiamo, soprattutto sulle questioni di tutela della salute e dell'ambiente, il federalismo e la

Il problema è presente anche per quanto riguarda lo Stato e il Governo.

perché tra le 8.500 imprese, come ovunque, ci sono i furbi e quelli che invece vogliono svolgere la loro professione con correttezza. utilizzano i filtri, che adottano tecniche produttive per ridurre l'impatto ambientale hanno maggiori costi e si troveranno di fronte a un'azienda, magari dall'altra parte della strada o in una città vicina,

implode. Una serietà, un richiamo o un afflato non si sentono. C'è la pratica o la pratichina da evadere e l'amico imprenditore da far passare.

niente. Se si va avanti così, è inutile che pretendiamo di mettere la parola ambiente, di differenziarci tra ambientalisti, AN, PD tratta di una marmellata dove nessuno ci capisce più niente. A rimetterci è il Paese. Cominciamo a fare le cose con serietà e a dare l'idea che abbiamo l'obiettivo di ridurre l'inquinamento e di premiare gli imprenditori seri.

il relatore e il Governo, pur riconoscendo l'assoluta inadeguatezza del termine del 31 marzo 2008 (l'ha riferito anche il rappresentante del Governo), non ritengono di dover prorogare

il mondo imprenditoriale italiano. Sono state fatte delle cifre: 8.500 imprese hanno avanzato le loro istanze e non hanno avuto ancora nessuna risposta. Mi dispiace che la senatrice De Petris interpreti il ruolo del Governo come quello di una piccola amministrazione locale ripartendo, secondo le competenze, la responsabilità. Governare è tutt'altra cosa. Governare un Paese è soprattutto avere una interfaccia diretta con la Comunità Europea, dinanzi alla quale abbiamo delle responsabilità che poi puntualmente si traducono in procedure di infrazione. Governare un Paese non significa vedere quanta percentuale di responsabilità abbia la Regione, una Provincia, un Comune o una circoscrizione, ma abbracciare l'intera responsabilità sul territorio nazionale che un Governo deve avere. Dagli interventi di esponenti della stessa maggioranza sono emerse perplessità evidenti sull'operato del Ministero dell'ambiente in questa materia come in tante altre. Io mi sono riferito anche ad altre materie, in via generale, nel mio intervento, perché se dovessi scendere nell'analisi delle inadempienze del Ministero dell'ambiente

enorme contesto di inefficienza che fa capo al Ministero dell'ambiente e che non ho difficoltà a ribadire anche in questa sede in cui trattiamo una materia specifica ma non avulsa dal contesto di una politica di protezione e di gestione dell'ambiente, che questo Governo sta dimostrando di non saper fare. Quindi non parteciperemo al voto nel rispetto di quelle aziende parteciperemo sicuramente, come abbiamo fatto sempre, alla discussione e al voto del prossimo provvedimento, inevitabile, quando al 31 marzo 2008 si dovrà, ancora una volta in zona Cesarini come si suol dire in termini sportivi, intervenire:

degli imprenditori ma per inefficienza dell'apparato pubblico; quelle 8.500 aziende si troveranno ancora una volta, nell'arco di 24 ore, a rischio di chiusura. Anche il fatto che un provvedimento di questo tipo si emani il giorno stesso in cui decadono i termini sta a dimostrare l'assoluta superficialità con cui il Governo pone attenzione ai fatti della produzione e del rispetto delle direttive comunitarie. Non è più tollerabile e io spero che il Governo non sia quello che dovrà proporre il prossimo differimento dei termini, perché se dovesse ancora essere in vita al 31 marzo 2008 il Paese sarebbe veramente completamente allo sfascio.

dall'altro, però, non possiamo non stigmatizzare in modo forte il fatto che neppure l'intelligente appello che era stato rivolto

Quindi, forti della consapevolezza che il ruolo delle imprese italiane deve essere difeso, ma parimenti consapevoli del fatto che vi è stata una fortissima miopia di atteggiamento

Non stiamo parlando di quelli nuovi, che hanno un percorso ordinario, ma di come dovevamo adeguare a questa nuova norma i circa 8.000 impianti disseminati sull'intero territorio nazionale. Si sarebbe quindi dovuto pensare - ed è questo il senso del nostro ordine del giorno - ad un modo di provvedere a queste autorizzazioni

Ciò non è ancora stato fatto e tale deve essere l'obiettivo che il Governo si deve porre nelle prossime settimane, prima del prossimo 31 marzo; questo è l'obiettivo che indichiamo nell'ordine del giorno. Vorrei che fosse chiaro a tutti in quest'Aula che stiamo esaminando un provvedimento che serve alle aziende per poter produrre e continuare la propria produzione nel quadro di compatibilità ambientale definito a livello europeo.

reca: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004ۚ». Il relatore, senatore Del Roio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Honduras, fatto a Tegucigalpa il 7 maggio 2004.

che riguarda principalmente la situazione dei diritti umani dei popoli indigeni in Honduras e in buona parte anche la situazione del popolo dei Garifuna, afrodiscendenti che sono oggi maggiormente "impattati" da progetti di sviluppo e da grandi infrastrutture del settore turistico

nel modo seguente: «ad esaminare con attenzione la possibilità di procedere alla ratifica della Convenzione ILO 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro»,

al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, è stata sottoscritta il 28 marzo 2006.

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero per il rinnovo della concessione relativa al collegamento della rete ferroviaria svizzera con la rete italiana attraverso il Sempione dal confine di Stato a Iselle e l'esercizio del tratto da Iselle a Domodossola, fatta a Torino il 28 marzo 2006*** Il disegno di legge oggi in esame è già stato approvato alla Camera il 17 luglio 2007 e ne prevede la ratifica, pur con un ritardo di diciotto in modo sintetico alcuni passaggi significativi. La precedente concessione era stata istituita dalla Convenzione del 22 febbraio del 1896 e aveva la durata di novantanove anni a partire dalla data di attivazione della linea ferroviaria, che risale al 1° giugno del 1906; pertanto, è scaduta il 31 maggio 2005.

L'oggetto della concessione è la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, ivi inclusa la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza connessi alla circolazione dei convogli e la progettazione, la realizzazione e la messa in esercizio delle nuove costruzioni e tecnologie, necessarie per l'adeguamento dell'infrastruttura ferroviaria alla disposizione normative e alle esigenze del traffico. Negli articoli 3 e 4 sono riportati gli obblighi del concessionario e le condizioni. All'articolo 5 si affronta il tema dell'esercizio tra Iselle e Domodossola e, in particolare, si precisa che i gestori dell'infrastruttura italiano e svizzero procederanno alla stipula di una convenzione che regoli le condizioni di esercizio e di prestazione di servizi che possono essere forniti reciprocamente in sinergia, relativamente alla tratta di confine tra Iselle e Domodossola. I gestori dell'infrastruttura potranno anche concordare tra loro, previa approvazione dei Governi, un'estensione territoriale della gestione unitaria della tratta ferroviaria. L'articolo 6 affronta il tema degli accordi collaterali (poste, dogane telecomunicazioni e servizi di polizia), gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 affrontano tematiche procedurali legate all'osservanza della sovranità o della difesa nazionale. In conclusione, in

sede di esame del disegno di legge 1726 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Città del Guatemala 1'8 settembre 2003»,

Presidente, onorevoli senatori, l'Accordo in esame è volto a realizzare un quadro giuridico di riferimento diretto a favorire e conferire garanzie agli investimenti allo scopo di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche e dell'interscambio commerciale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Guatemala. In particolare, esso si colloca nell'ambito degli accordi in materia che l'Italia e gli altri Paesi dell'Unione Europea hanno, negli ultimi anni, firmato con vari Paesi dell'area al fine di incoraggiare, in un quadro di maggiori certezze e più precise garanzie, ulteriori iniziative imprenditoriali e un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle Parti contraenti. Nel merito, all'articolo 1 l'Accordo definisce in maniera ampia il termine "investimento", soprattutto in relazione alla necessità di includere il maggior numero possibile di attività economiche nel meccanismo di tutela ivi previsto. L'articolo 2, nell'ambito dell'obiettivo sopra descritto, di promozione e protezione degli investimenti, stabilisce l'obbligo di garantire un diritto di accesso alle attività di investimento non meno favorevole di quello assicurato ai propri cittadini articolo 3), nonché di assicurare un trattamento "giusto ed equo" agli investimenti degli investitori di ciascuna Parte nei loro reciproci territori. Al riguardo, il successivo articolo 3, nel prevedere l'applicazione di un trattamento giuridico pari a quello concesso agli investimenti e ai redditi ricavati da propri cittadini o da cittadini di Stati

L'articolo 5 interviene in tema di nazionalizzazioni, espropriazioni o misure analoghe, precisando che non potranno avvenire direttamente o indirettamente se non per motivi di ordine pubblico o per interesse nazionale, su base non discriminatoria. Si rileva la norma di cui all'articolo 7, volta a tutelare gli organismi di assicurazione degli investimenti, che prevede il diritto di surroga di tali organismi nell'esercizio dei diritti e nelle pretese dell'investitore nei casi di risarcimento per danni o perdite. All'articolo 9 dell'Accordo si prevede che, in caso di controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell'altra parte contraente, in primo luogo si dovrà cercare di comporre tale controversia in via amichevole entro sei mesi. All'articolo 11 si stabilisce che l'esecuzione dell'Accordo sia assicurata a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le due Parti.

l'entrata in vigore e la durata del medesimo. Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli, rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge. In conclusione, si propone di approvare il disegno di legge e di procedere alla ratifica del documento.

a nostro parere, stanno aprendo una nuova fase, una nuova stagione in un Paese martoriato per anni da dittature e violazioni dei diritti umani dei popoli indigeni. L'ordine del giorno vuole far tesoro di questa opportunità richiamando alcune recenti denunce di *Amnesty International* e di altre organizzazioni internazionali per i diritti umani relative alle persecuzioni degli attivisti

si chiede un impegno forte del Governo italiano affinché vengano affrontate tali questioni nei rapporti bilaterali e venga sostenuta la creazione di una Commissione internazionale di inchiesta contro l'impunità in Guatemala a nostro parere un elemento fondamentale per costruire le premesse per una nuova democrazia. Inoltre, si invitano le imprese italiane che operano in Guatemala al rispetto dei diritti dei popoli indigeni e delle norme fondamentali del lavoro. Vorrei richiamare un unico esempio, con riferimento ad un investimento italiano nel municipio di Chajul per la costruzione di una diga sul fiume Jute, un'infrastruttura che rischia di impattare negativamente sulle condizioni di vita delle popolazioni indigene locali. Si immagina che qualsiasi investimento in quel Paese, come del resto anche in altri Paesi,

***Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali,

Presidente, onorevoli senatori, l'Accordo in esame sostituisce quello precedente concluso con l'Argentina in tema di coproduzione cinematografica, firmato a Roma il 9 dicembre 1987 e ratificato ai sensi della legge n. 306 del 1989. Esso aveva già tracciato un quadro normativo di riferimento nella prospettiva dello sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi e ora viene aggiornato con modifiche ritenute necessarie alla luce dell'applicazione del citato Accordo e del mutato contesto normativo internazionale, soprattutto a livello comunitario. In particolare, tra le principali innovazioni si segnala che all'articolo 1 in primo luogo, il significato di coproduzione cinematografica in termini più estensivi rispetto alla precedente formulazione, tenendo conto dei progressi tecnologici intervenuti nel settore; individua altresì, quale autorità competente dell'applicazione dell'accordo per l'Italia, il Ministero per i beni e le attività culturali (Direzione generale per il cinema). I successivi articoli 2 e 3 confermano i principali contenuti della attività di coproduzione, stabilendo che i film coprodotti, una volta ricevuta l'approvazione da parte delle competenti autorità nazionali, godono degli stessi vantaggi dei film nazionali, ove realizzati da imprese che posseggono una buona organizzazione tecnica ed una riconosciuta reputazione professionale. Si confermano inoltre le disposizioni in tema di produzioni multilaterali con Paesi con cui una delle parti ha sottoscritto accordi di coproduzione (articolo 6); di possesso del negativo originale da parte di entrambi i coproduttori (articolo 7); di ripartizione dei proventi tra i coproduttori corrispondenti alla percentuale rispettivi apporti; di presentazione di film con la dicitura coproduzione italo‑argentina ovvero coproduzione argentino-italiana, nonché infine di partecipazione ai festival internazionali da parte del coproduttore maggioritario. Si detta infine una disciplina dettagliata rispetto alla precedente formulazione circa le funzioni della commissione mista che, oltre al riconoscimento del potere di proposta di eventuale modifica dell'accordo da sottoporre alle rispettive autorità di Governo, è altresì competente ad esaminare l'equilibrio complessivo delle coproduzioni in relazione al numero delle stesse, all'ammontare degli investimenti e agli apporti partecipativi. Il disegno di legge, infine, si compone di 4 articoli concernenti l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le norme di copertura finanziaria e l'entrata in vigore. Alla luce delle suddette considerazioni, si propone di approvare il disegno di legge e di procedere alla ratifica del documento.

Come dire che i simboli della comunità internazionale sono indicati da Al Qaeda come simboli del nemico nei confronti del radicalismo islamico, al di là e al di fuori di interventi occidentali o di presenza di eserciti a Baghdad e non ad Algeri.

Signor Presidente, ringrazio il relatore Mantica, perché la ratifica del trattato con l'Algeria offre l'occasione per richiamare l'attenzione dell'Aula su quanto accaduto ieri nella capitale di uno Stato che dista poche decine di miglia miglia dai nostri confini meridionali. È un'attenzione che ritengo non solo doverosa, ma anche necessaria, dal momento che gli attentati e forse lo dimostra anche l'attenzione con cui queste povere parole vengono accolte in questo momento - sembrano avere una gravità inversamente proporzionale rispetto all'eco che stanno avendo da noi. Da noi ci si occupa di questioni certamente più importanti, dai capricci del Ministro della giustizia alla quota proporzionale o maggioritaria di un ipotetico sistema elettorale, ma per chi abbia voglia di interessarsi della vicenda gli elementi di preoccupazione sono tanti e pesanti: 67 morti, tra cui circa 20 giovani universitari e una decina di funzionari dell'ONU; un centinaio di feriti; 13 dispersi; il numero del giorno scelto per la tragedia, torna il simbolo 11

Gli obiettivi: la sede del Consiglio costituzionale algerino, la sede dell'Alto consiglio islamico e, come già ricordava il relatore, la sede dell'Alto commissariato ONU per i rifugiati, con un sinistro rinvio a quanto accaduto nell'agosto del 2003 a Baghdad. Da ultimo, ma non in ordine logico, la rivendicazione di Al Qaeda in Marocco, in continuità con la minaccia rappresentata in passato dal gruppo salafita per la predicazione e il combattimento. Presidente, l'Algeria non è un Paese occidentale né, a differenza di altri Stati a maggioranza islamica, si mostra particolarmente vicino all'Occidente, visto che da anni è tra i capofila dei cosiddetti non allineati. Dunque, per l'ennesima volta, gli attentati non rappresentano la reazione ad una presunta oppressione americana o occidentale, ma lo strumento politico tragico per richiamare all'unità dell'Islam in un'ottica ultrafondamentalista. Nessuna riserva ovviamente sul trattato in discussione, ma il Governo italiano, oggi presente attraverso il Vice Ministro degli esteri, ha il dovere di rendere un'informativa completa rispetto a quanto è accaduto; di aggiornare sul livello di collaborazione, non soltanto giudiziaria, che è oggetto di questo trattato, ma, in senso lato, di polizia e tra servizi; di chiarire quali sono i livelli di rischio per la nostra Nazione derivanti da attentati che si svolgono ai confini meridionali di casa nostra e quindi qual è il tipo di attività di prevenzione che oggi viene svolto su questo fronte.

dal punto di vista dei diritti umani e della preoccupazione per questo terrorismo che continua ad essere una sfida al fianco dell'Occidente, così come di alcune regioni islamiche. Ricordiamo che il primo obiettivo del terrorismo islamico sono quei Paesi islamici che mantengono - lo ha ricordato il collega - seppure con difficoltà un rapporto di dialogo con l'Occidente e un sistema quanto meno democratico o che non ceda alle sirene del fondamentalismo. C'è un mondo di dissidenti, come abbiamo visto anche in questi giorni, che sta pagando con la pelle il tentativo, al pari di Sakharov in Russia, di costituire in questi Paesi un baluardo di democrazia. Credo che questo appello non possa rimanere inascoltato anche dal Parlamento, che questo attentato contro l'Alto commissariato per i rifugiati, contro le istituzioni,

Onorevoli senatori, alla notizia dell'attentato sanguinoso, drammatico di ieri che ha colpito le strade di Algeri il Governo non ha esitato un secondo a a dichiararlo infame, soprattutto se si considera l'amicizia tra il popolo italiano e quello algerino e, ancor di più, l'impegno che abbiamo assunto la scorsa settimana in occasione della visita del presidente Bouteflika non soltanto in materia di cooperazione economica, ma soprattutto in materia di cooperazione giudiziaria e di sicurezza per i nostri Stati; cooperazione giudiziaria, tra l'altro, inerente al al Trattato che stiamo ratificando. Sul piano della sicurezza più in generale è evidente che il recente allarme lanciato il recente allarme lanciato in merito alla presenza di gruppi salafiti armati in tutta la cintura del Maghreb vede in prima fila i Paesi coinvolti, ma anche le nostre forze di sicurezza che, non a caso, hanno stipulato con le analoghe forze di sicurezza algerine dei Paesi del Maghreb accordi di cooperazione. Non sono sufficienti l'indignazione, sufficienti l'indignazione, il nostro cordoglio e la nostra commozione, pure alti. Alta deve essere anche la nostra guardia e il nostro senso di cooperazione politica, giudiziaria, militare e di polizia.

una gestione integrata paneuropea del traffico aereo. Essa quindi sviluppa coordina e pianifica le strategie di controllo del traffico aereo, a breve e lungo termine, coinvolgendo nel processo autorità nazionali, fornitori di servizi, utenti civili e militari, aeroporti, industrie, organizzazioni professionali ed altre istituzioni europee rilevanti. Per quanto riguarda i contenuti di questi due

122 milioni di unità nel 2006. Il numero di tonnellate movimentate è passato da circa 655.000 unità nel 1996 a circa 911.000 unità del 2006. Nel 1960, anno della firma della prima convenzione, l'Unione Europea era composta da soli cinque Stati; oggi siamo ormai di fronte a 27 Stati membri. Nel 1960 e fino al 1989 eravamo ancora in presenza di due blocchi contrapposti, che non avevano accettato nessuna iniziativa comune in merito alla sicurezza degli aeromobili; oggi siamo finalmente di fronte ad un codice comportamentale che consente ad un singolo Stato di bloccare, se lo desidera, una compagnia aerea qualora non corrisponda a determinati requisiti. Nel 1960 nessuno pensava a forme innovative, come il sistema GPS o come quello definito dal progetto Galileo; oggi siamo ormai vicini alla costruzione di un sistema - quello definito proprio dal progetto Galileo - al servizio di tutti i Paesi europei. Il *low cost*, l'ottimizzazione delle procedure di avvicinamento agli scali aeroportuali, il contenimento dei costi energetici e la logica degli *hub* sono tutte aree tematiche strategiche che vengono condivise all'interno di un teatro economico internazionale;

oltre a far conseguire dei benefici per i settori industriali e commerciali interessati, può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi e allo sviluppo degli interscambi, in maniera da sviluppare uno spirito di amicizia che del resto è già esistente. Esso potrà anche contribuire

con ricorso del 12 giugno 2007, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 30 gennaio 2007, ha dichiarato che i fatti oggetto n. 6259/03 RG GIP, pendente nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi, concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 19 novembre 2007, n. 399, depositata in cancelleria il successivo 23 novembre. La questione se il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in data 4 dicembre 2007. Nella seduta di ieri la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso, a maggioranza, in senso favorevole alla costituzione in giudizio. Se l'Assemblea converrà con le conclusioni cui è pervenuta la Giunta, la Presidenza si intenderà autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro. Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

al Senato di costituirsi nei giudizi davanti alla Corte costituzionale. Dicevo, come premessa, che il fatto è particolarmente grave perché il figlio e il coniuge di un sindacalista UIL, ucciso nell'ottobre del 1998, con una querela si erano lamentati e avevano segnalato che sul loro congiunto era stato scritto, all'interno di un articolo di "Panorama", a firma dell'attuale senatore Iannuzzi, che un sindacalista, appunto Domenico Geraci che era molto discusso, avrebbe fatto da tramite tra la mafia e ambienti di sinistra. Nella querela veniva segnalata e rivendicata una posizione di costante contrasto nei confronti della mafia in molteplici settori dell'attività economica, politica e amministrativa dei mafiosi e dei criminali appartenenti ad una associazione che veniva contestata come criminosa. Sul fatto credo si dilungherà il senatore Larizza, all'epoca segretario generale della UIL.

Ricordo che il 30 gennaio 2007 il Senato, a maggioranza, ha ritenuto di non dover concedere l'autorizzazione a procedere per il grave fatto che ho segnalato e, come era scontato peraltro, il GIP di Milano aveva sollevato conflitto di attribuzione con il Senato davanti alla Corte costituzionale proprio perché riteneva infondata e gravemente lesiva delle prerogative costituzionali quella decisione del Senato. Come altrettanto scontato, la Corte costituzionale ha ammesso il conflitto sollevato dall'autorità giudiziaria di Milano e, a questo punto, il Senato si trova a dover decidere su una questione che è solo in apparenza formale, cioè deve decidere se sostenere e difendersi Il problema è: da che cosa deve difendersi? Questo ci porta al motivo per cui, all'interno della Giunta, i membri del Gruppo si sono espressi o contro o per l'astensione e comunque, al momento del voto, si sono tutti astenuti.

perché in questa situazione la Corte costituzionale, per sua giurisprudenza pressoché costante in questi ultimi anni, ha ritenuto di dare torto alla posizione del Senato.

altrimenti non ci sarebbe la previsione della necessità di una nuova autorizzazione. Di fronte a una posizione che riteniamo perdente e sbagliata, proprio per il comportamento e per la giurisprudenza della Corte costituzionale, rappresento che in questa causa, che non ho dubbi a definire persa, si verrebbe a costringere il Senato ad ulteriori spese rilevanti da affrontare per il giudizio e per gli avvocati. In conclusione, ritengo che non possa essere espresso un voto favorevole alla richiesta di costituzione in giudizio davanti alla Corte costituzionale.

perché esso rimane assorbito nella decisione che la Giunta ha consacrato con la sua deliberazione. È giusto in quella sede sostenere tesi contrarie, dire di non essere d'accordo e, ancora di più, il merito rimane cristallizzato nella decisione finale che poi quest'Aula ha assunto. È chiaro che io in quel contesto avrei anche potuto essere contrario alle tesi che sostenevano altri, ma quando quelle tesi diventano patrimonio comune perché l'unico consesso democratico deputato a decidere è quest'Aula, alla fine, applicando una regola democratica, quella del voto della maggioranza e dell'opposizione, e decidendo che la volontà del Senato è rappresentata da quella indicazione, per me essa nel merito non diventa più contestabile. È come se io

perché l'oggetto della decisione che viene sottoposta all'Aula in questo momento è assolutamente un altro. La Giunta decide, l'Aula decide e quindi un organo dello Stato, il Parlamento, decide di esercitare in un certo modo una sua funzione e una sua attribuzione che discende direttamente dall'articolo 68 della Costituzione. Nel nostro ordinamento è previsto il conflitto di attribuzione fra organi dello Stato proprio perché un organo dello Stato possa chiedere alla Corte costituzionale se nella valutazione di una determinata situazione un altro organo abbia abbia travalicato i limiti che la Costituzione pone. Ora siamo esattamente in questa situazione: infatti, il tribunale di Milano impugna la deliberazione assunta dal Senato davanti alla Corte costituzionale alla quale chiede di valutare se la delibera assunta dal Senato rientri nei limiti costituzionali di cui all'articolo 68 o meno. Siamo in una sede di conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato rispetto alla quale la Corte costituzionale, in via preliminare, si riunisce e decide che il conflitto è astrattamente ammissibile. Signor Presidente, rispetto a questa situazione dobbiamo solo decidere se il Senato abbia diritto di difendere le sue ragioni oppure no e io non capisco perché dobbiamo essere tutti pronti a scagliarci contro coloro i quali vogliono limitare il diritto di difesa riconosciuto dalla nostra Costituzione in favore di tutti ed invece in questa sede non vogliamo riconoscere il diritto di difesa al Senato della Repubblica. Posso non condividere nel merito le cose che il Senato ha avallato in Aula, posso anche averle contestate, però le regole democratiche ci impongono poi di rispettare rispettare la volontà legittimamente assunta dal Senato, anche quando quella volontà non la condividiamo, anche quando quella decisione l'abbiamo avversata. L'oggetto della valutazione alla quale oggi siamo chiamati non è il comportamento del senatore Iannuzzi nel momento in cui scriveva l'articolo, non è la legittimità delle pretese degli eredi, della moglie e del figlio, del sindacalista della UIL: purtroppo non è questo, perché questo merito è già coperto dal giudicato che in qualche modo l'Aula del Senato ha formato.

merito siamo stati tutti contrari, ma ciò non cambia il senso della vicenda che viene sottoposta al nostro esame. Siamo di fronte ad un diritto secondo me indisponibile. Dico anche perché (ed affronto il merito in maniera molto larga) in questo caso il tribunale di Milano ha riconosciuto che la Giunta e poi hanno ritenuto che il comportamento del senatore Iannuzzi fosse coperto dall'articolo 68 della Costituzione perché c'erano delle cose che nell'esercizio della funzione il senatore Iannuzzi aveva fatto (due disegni di legge in materia di mafia che in qualche modo richiamavano l'argomento), però lo stesso tribunale ha rilevato che non c'è quella perfetta coincidenza che la Corte costituzionale reclama per rendere operativo l'articolo 68. Siamo cioè in una fase nella quale il merito largo, non il merito pieno, oggetto della contestazione del tribunale di Milano, che solleva conflitto di attribuzione, in qualche modo merita di essere difeso, la tipicità della funzione parlamentare che tutti esercitiamo a volte viene resa più labile anche da alcuni strumenti parlamentari. Vale a dire che quando la Corte pretende che ci sia perfetta coincidenza tra le cose che il parlamentare dice dentro il Parlamento nell'esercizio della funzione e le cose che dice fuori, non considera che in alcuni casi

coincidenza integrale che la Corte pretende. Ed allora, in questo caso, cosa succede? Che le cose che il parlamentare ha detto nell'esercizio della funzione non in Aula, ma in Commissione di merito,

potrebbe dare luogo a vicende assolutamente antipatiche. Infatti, se il senatore Iannuzzi avesse voluto precostituirsi una insindacabilità assoluta,

ci sono delle valutazioni che vorrei la difesa del Senato cominciasse a prospettare alla Corte, e questo è possibile se c'è una difesa, un esercizio di un diritto che viene consentito a questa Assemblea. Concludendo, non ho condiviso il merito della decisione assunta dall'Assemblea. Ritengo, però, che la decisione vada rispettata e che il Senato debba essere autorizzato a costituirsi per coltivare quel diritto alla difesa che insieme all'Assemblea difenda l'istituzione e tutti quanti noi, anche quelli che la pensano diversamente.

del senatore Manzione e devo dire che nel confronto quelle che mi hanno convinto di più e meglio sono quelle del collega Manzione, che pone un tema di carattere generale. Mi meraviglio che il collega Casson abbia pensato ad una rivalutazione, ad una "respirazione artificiale" del merito, quando invece qui dobbiamo stabilire un equilibrio che riguarda, tra i poteri dello Stato, quello che, avendo svolto una funzione critica rispetto alla posizione assunta dal Senato, ha posto la Corte costituzionale in grado di decidere se debba prevalere la decisione di quest'Aula

una specie di esercitazione di pronostico. Il pronostico, se è giusto o non è giusto, lasciamolo decidere a quelli che nelle valutazioni di carattere giudiziario si comportano qualche volta come dal barbiere «Bella Napoli». Credo, invece, che la Corte costituzionale debba decidere la sussistenza o no di un potere autonomo e autogeno, che è quello del Senato della Repubblica, di assumere, di fronte all'atteggiamento di un senatore, un rapporto che è stato già formalizzato e deciso in termini di coerenza. Coerenza vuole che la decisione sia difesa, coerenza vuole che davanti alla Corte costituzionale si pongano i problemi nelle condizioni di parità, con le diversità di valutazioni e con la funzione dialettica e la diversità consenta al giudice di stabilire, futura sua sintesi non pronosticata ma valutata nel concreto, che cosa si debba fare o no. Difendere le proprie posizioni mi pare sia

Nell'articolo di "Panorama" era scritto, tra l'altro: «un sindacalista molto discusso, che avrebbe fatto da tramite tra la mafia ed ambienti di sinistra

Dopo la sua morte sono andato a Caccamo per un'iniziativa unitaria organizzata dal sindacato, cui erano presenti non solo tutte le autorità dello Stato e della Regione, ma anche tutte le forze sociali del lavoro e dell'impresa, non solo per condannare il fatto ma per confermare la lotta intransigente contro la criminalità organizzata e la mafia e per riconoscere proprio a Geraci il titolo di sindacalista onesto e perbene che, in quanto tale, aveva pagato con la vita questo comportamento. Caccamo, il paese in cui è stato ucciso, non a caso era chiamato la Svizzera della Sicilia, perché sotto il controllo ferreo della mafia, il cui capo mandamento era Giuffrè, ora un pentito. Geraci era uno fra i pochissimi che contestava quella gestione, che contestava l'amministrazione, che dava fastidio ad una gestione di mafia che blindava un paese intero. Questo era Geraci!

che non solo era una persona perbene, ma che i carabinieri avrebbero fatto, come al solito, il loro dovere ed anche qualcosa in più per catturare gli assassini. allora, è un'occasione non per discutere le formule tecniche e giuridiche, sulle quali siete tutti più esperti di me, ma per fare un punto di verità fondamentale, che tra l'altro dà forza al mio voto in dissenso. Quella figura, la figura del sindacalista Domenico Geraci, è stata esemplare per il mondo del lavoro italiano e per la Sicilia.

determinazione che ha condotto alla dichiarazione di insindacabilità del senatore Iannuzzi nel procedimento contro di lui aperto davanti al tribunale di Milano. Noi, invece, siamo assolutamente d'accordo e assolutamente convinti della bontà di quella scelta

se il senatore Iannuzzi debba o meno essere dichiarato portatore di insindacabilità con riferimento alle cose dette e, quindi, sottratto al procedimento penale. Oggi il tema in discussione è se il Senato si debba o meno costituire davanti all'organo di giustizia che, a legge vigente, deve deve pronunciarsi su un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato legittimamente dal tribunale di Milano. Sull'opportunità altro si potrebbe dire, ma sulla legittimità nulla può essere revocato in dubbio. Noi siamo convinti che il Senato debba costituirsi in giudizio in questa e in ogni altra occasione e quindi il voto che preannuncio a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale è favorevole.

con l'ordine del giorno che sarà deliberato dalla Conferenza del Presidenti dei Gruppi parlamentari convocata per le ore 12,15. La seduta è tolta